seduta è tolta *(ore 13,20)*. *Allegato A* DISEGNO DI LEGGE Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

onorevoli colleghi, ho ascoltato con grande attenzione gli interventi che si sono succeduti nel corso del dibattito di ieri,

hanno concordato su un dato - che appartiene peraltro alla pubblica cognizione, non bisogna certamente fare particolari sforzi per avere conoscenza di ciò che la giustizia in Italia costituisce un problema non secondario, che la giustizia in Italia non dà le risposte che dovrebbe dare, che la giustizia italiana è particolarmente lenta, che in Italia tanto bisogna fare per ripianare i disagi che questo tipo di giustizia determina. Signora Presidente, ho ascoltato con particolare attenzione il suo intervento e ho preso nota delle sue considerazioni, che condivido quasi integralmente. Condivido certamente la diagnosi, condivido le valutazioni, non condivido alcune sue conclusioni, perché ritengo che, a volte, talune occasioni contingenti forniscano la possibilità di intervenire per risolvere problemi annosi e che chi ha la responsabilità di risolverli non si possa sottrarre, al di là delle ragioni che determinano questi interventi.

fatto da chi conosce, e non da oggi, quali sono i problemi della giustizia, la loro entità. quel caso ho ascoltato critiche - critiche serrate, portate con piena cognizione - ma non ho ascoltato proposte.

archi temporali assolutamente irrilevanti rispetto all'ampiezza dei termini che sono effettivamente previsti per la celebrazione dei processi e, in particolare, sarebbero molto più contenuti rispetto a quelli che noi abbiamo previsto con questo disegno di legge.

L'articolo 111 ci impone di intervenire. Ieri è stato rammentato dal collega Mazzatorta che anche un autorevole organismo internazionale, la Commissione europea nel momento in cui ipotizzava un Programma quadro per tutti i Paesi dell'Unione europea, li invitava ad intervenire per definire anticipatamente la durata dei processi. rivolgere critiche a questo disegno di legge assolutamente immotivate. Qualcuno, con argomenti che hanno sempre intrinsecamente una loro suggestione, perché la tematica che trattano coinvolge e naturalmente viene viene sempre ascoltata con particolare attenzione, ha detto che abbiamo previsto tempi ragionevoli anche per la mafia: abbiamo previsto tempi ragionevoli per i processi di mafia e di terrorismo, come era nostro dovere, nel rispetto del precetto costituzionale.

Lo abbiamo fatto perché era nostro dovere e lo abbiamo fatto tenendo conto delle esigenze che quei processi comportano. Non sono processi che si possono esaurire in poche battute: impegnano il giudice in una valutazione complessa perché una messe di elementi e documenti viene sottoposta al suo giudizio. Allora, abbiamo ipotizzato dei tempi assolutamente congrui e coerenti. La ragionevole durata, signora Presidente, deve essere il punto di equilibrio fra il contenimento temporale del processo e l'esigenza effettiva della giurisdizione: questo è il giusto processo. Non basta dire che i tempi devono essere brevi: è la capacità di individuare una sintesi fra esigenze complesse e e la conclusione del processo. Questo sforzo ci siamo impegnati a realizzare. Mi consenta una considerazione, signora Presidente. Nel corso degli ultimi dieci anni abbiamo istituito giudici nuovi, sia pure onorari. Intorno al 1998 - chiedo venia se non rammento le date con precisione - per consentire lo smaltimento dei cosiddetti processi stralcio del civile, quelli cioè trattati con il vecchio codice di procedura civile,

rito dovesse poi anche impaludarsi nelle vicende dei processi trattati con il rito precedente. Ma soprattutto lo spirito fu quello di sottrarre alla giurisdizione onoraria 5 milioni di processi che dovevano essere conclusi egualmente. I GOT hanno assunto la cognizione di questi processi e quindi, alla metà degli anni '90, 5 milioni di processi vengono sottratti alla giurisdizione che chiamiamo con espressione impropria La figura del giudice di pace assume una nuova connotazione: oltre ad occuparsi di vicende civili, si occupa anche di vicende penali. Guardate quanti interventi vengono fatti per ottenere l'obiettivo principe di una giurisdizione di un Paese civile con una grande tradizione giuridica come la nostra. Anche il giudice di pace è investito della cognizione di un numero sensibile di processi che vengono sottratti alla giurisdizione professionale. Eppure, arriviamo nel 2010 e siamo costretti ad ascoltare le cifre che ieri sono state indicate dal presidente Berselli per documentare in termini inequivoci ed indubitabili la tragicità della situazione dei processi nel nostro Paese. Allora, abbiamo l'obbligo di scrivere le regole. Poi ognuno degli operatori della giustizia - siano essi avvocati, funzionari, magistrati - assumerà la responsabilità della nuova condizione. assumerà la responsabilità della nuova condizione. Certamente i tempi che sono stati previsti non sono tanto contenuti da non poter consentire, se non con frenetica attività, la risoluzione delle vicende processuali nelle quali sono impegnati. Signora Presidente, mi avvio alla conclusione, confidando che l'Assemblea comprenda, al di là della della dialettica che è fisiologica e delle contrapposizioni che sono il sale della democrazia, quali sono le ragioni reali...

hanno indotto finalmente il legislatore ad assumere l'iniziativa della quale in questi giorni dovremo discutere e che io mi auguro vivamente diventi legge dello Stato. *(Applausi

Signora Presidente, abbiamo assistito in questi giorni, nell'attività del Senato, sia in sede di Commissione giustizia che in Aula, ad una trasformazione per così dire camaleontica di un disegno di legge che era stato presentato come misura indispensabile per salvare il processo (in particolare penale) in Italia. Veniva indicato come il toccasana. Dall'inizio questa maggioranza e questo Governo parlavano del processo breve, soprattutto a livello di opinione pubblica, come soluzione della grave piaga dei tempi processuali che colpisce il nostro sistema giudiziario. Ora, di fronte al problema che esiste e che è gravissimo (diciamo pure che è vergognoso), viene proposta una misura che di fatto aveva e ha tutt'altri effetti rispetto a quelli necessari al nostro sistema processuale, in particolare penale. sappiamo benissimo come nasce questo disegno di legge, sappiamo benissimo quali sono le sue finalità e sappiamo benissimo come, nonostante la trasformazione camaleontica di alcune di queste norme, il fine ultimo, cioè quello di salvare il Presidente del Consiglio dei ministri, sia rimasto intatto ed evidentissimo in tutti i suoi aspetti negativi, con particolare riferimento al profilo della legittimità costituzionale. Vediamo cosa è successo in questi giorni di esame del disegno di legge. Non a caso, forse, quasi per un *lapsus* freudiano, il titolo del disegno di legge recitava "misure per la tutela del cittadino" (aggiungeremmo: del cittadino Berlusconi). Subito sono emersi evidenti problemi di legittimità costituzionale, profili di legittimità costituzionale che non potevano essere assolutamente dimenticati da alcuno, ed erano talmente evidenti che perfino dai banchi della stessa maggioranza, all'interno in particolare della Commissione affari costituzionali, si sono levate delle osservazioni in senso contrario a sottolineare quelli che erano gli aspetti più gravi, che addirittura non avrebbero consentito al Presidente della Repubblica di promulgare una legge del genere, talmente palesi ed evidenti erano questi vizi, tanto più che di fatto non risolvevano il problema della celerità dei tempi processuali. Accanto a questi evidenti profili di illegittimità costituzionale, emergevano evidenti problemi di ragionevolezza nell'uso che veniva fatto delle norme, innanzitutto in relazione alla legge Pinto (alla procedura necessaria

con alcune norme che riguardavano il cosiddetto scudo fiscale. Di fronte a questi problemi evidenti, sono emersi anche i rischi fortissimi e pesanti di intralcio al sistema giudiziario nel suo complesso, a quella che definirei sinteticamente come macchina giudiziaria. Questo problema è stato segnalato già nelle fasi preliminari in Commissione giustizia grazie all'intervento, nel corso delle audizioni, dei membri non soltanto dell'Associazione nazionale magistrati ma, in particolare, del Consiglio superiore della magistratura e dei rappresentanti dell'avvocatura. Praticamente, tutte le categorie aventi a che fare con questo disegno di legge in contrasto durissimo con un provvedimento che crea soltanto intralci alla macchina giudiziaria. Si è anche discusso del numero dei processi che rischiavano di finire al macero,

e di avviso ai difensori, sempre peraltro nel rispetto del diritto della difesa, che continuiamo a ritenere un diritto fondamentale. Ora che il Governo e la maggioranza si sono resi conto che non aveva più senso, dopo le trasformazioni avvenute nel passaggio dalla Commissione all'Aula, continuare a parlare di processo breve, perché si sarebbero resi ridicoli, ecco che cercano di recuperare dicendo che di processo breve il Governo non ha mai parlato e che era una cosa inventata dai giornalisti. Si fa quindi richiamo a quello che è un sacrosanto principio costituzionale e di diritto internazionale costituzionalizzato che prevede la durata ragionevole del processo. Questo cambiamento è avvenuto con gli emendamenti presentati dal relatore direttamente in Aula. Ma per quale motivo, e che cosa è cambiato? Ovviamente, il relatore si è reso conto della insostenibilità dell'impostazione che era stata data dal Governo e dalla maggioranza a questo disegno di legge, ma si è altresì reso conto che doveva garantire il fine ultimo dello stesso, e cioè salvare in particolare una persona dai suoi processi. Quindi, ferma rimanendo Colleghi, per cortesia, intorno al resto, nel tentativo di parare il colpo e di presentare anche all'opinione pubblica, non solo al Parlamento, qualcosa che fosse minimamente presentabile ed accettabile. del Partito Democratico, non siamo assolutamente convinti che il tentativo sia riuscito perché, se alcuni vizi palesi, gravissimi e fondatissimi di legittimità costituzionale sono stati sanati, rimangono certamente altri vizi di legittimità costituzionale, che abbiamo già segnalato in quest'Aula

Innanzitutto, la questione fondamentale per la maggioranza è aver creato una nuova causa di estinzione del processo nel caso in cui le singole fasi non si concludano nei termini fissati da quello che viene indicato come

di una prescrizione processuale, destinata ad affiancare la prescrizione quale causa di estinzione dei reati, ai sensi dell'articolo 157

perché tale tentativo di modificare la legislazione in questa materia continuerà a produrre effetti permanenti, per sempre.

fino a quando non verrà ridimensionata o comunque modificata grazie ad interventi istituzionali, o del Parlamento o della Corte costituzionale. Su questa vicenda abbiamo chiesto al Governo di farci

ci trova assolutamente d'accordo, ma così come viene fatto dal Governo non può dare fondamento costituzionale all'estinzione del procedimento per decorrenza dei termini massima. Il requisito della ragionevolezza, infatti, è incompatibile con termini temporali perentori che non abbiano riferimento alla natura del reato, alla complessità e alla specificità dell'accertamento richiesto in concreto. Nella fase preliminare ho detto che si tratta di un principio costituzionalizzato, di un principio del diritto internazionale recepito dal nostro ordinamento. Qui ricordo che la stessa Corte costituzionale, nell'interpretare le disposizioni dell'articolo 111 della Costituzione, tante volte richiamato dalla maggioranza e dal Governo, ha rilevato che il principio della ragionevole durata deve essere considerato in rapporto alle esigenze di tutela di altri interessi costituzionalmente protetti che vengono in rilievo nel processo penale. Il diritto alla ragionevole durata del processo viene viene consacrato nell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed era stato consacrato ancora prima dagli articoli 24 e 111 della nostra Costituzione. Esso consiste

sono assolutamente inaccettabili e cozzano, come accennavo, con i princìpi della nostra Carta costituzionale. Ne citerò alcuni, perché se n'è discusso in quest'Aula anche ieri sera durante gli interventi in sede di dibattito. Proviamo a pensare alla questione dell'irragionevole assimilazione all'interno di ciascuna fascia di reati di fattispecie dal disvalore penale assolutamente diverso. D'altra parte, è stata proprio la Corte europea dei diritti dell'uomo che, valutando il principio della durata ragionevole del processo, è ricorsa a parametri quali, appunto, la natura del reato, la complessità degli accertamenti, la complessità di un giudizio, oltre alla necessità di valutare la condotta processuale della parte e ovviamente la condotta anche delle parti autorità procedenti, Quindi, suscita perplessità, ad esempio, l'esclusione dal novero dei reati di seconda fascia - che richiedono un approfondimento

quali quelli che derivano dagli infortuni sul lavoro, che derivano dalle malattie professionali, che derivano da fatti di circolazione stradale. E guardate che in questi giorni abbiamo avuto richieste e sollecitazioni di chiarimenti da tutte le Regioni d'Italia

siamo particolarmente sensibili (noi per ovvi motivi istituzionali e costituzionali), mentre c'è una sensibilità che appare diversa e di segno opposto della maggioranza, e del Governo in particolare. Si tratta dei reati che concernono i fatti di corruzione. L'esclusione del reato di corruzione dalla fascia alta per cui i termini di prescrizione sono più lunghi contrasta, oltre che con la sensibilità

gravissimo, che è quello di contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Anche di fronte alla richiesta che abbiamo rivolto al Governo di riferire dove sono le risorse finanziarie

a sanare questo vizio: ci è stato detto di no in sede di Commissione; vedremo se in Aula vi saranno dei ripensamenti. Comunque, c'è stato soltanto un rendersi conto della fondatezza della nostra osservazione, tanto è vero che un emendamento del relatore prevede che, di fronte ai problemi di ordine finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze

l'incendio; le lesioni personali anche aggravate; alcuni casi di mutilazione genitale; la distribuzione, cessione e detenzione di materiale pedopornografico; il sequestro di persona semplice; *stalking*; il furto nelle sue varie forme anche aggravate (poi vedremo cosa diranno i senatori della Lega nei loro territori quando sosterranno che loro tutelano i cittadini); la circonvenzione di incapace; molte violazioni delle norme contro gli infortuni sul lavoro; traffico illecito di rifiuti (tra l'altro, spesso il traffico illecito di rifiuti è un reato presupposto delle associazioni mafiose). Arrivo a quello che è il punto fondamentale di questo disegno di legge per il Governo e per la sua maggioranza: la disciplina transitoria. Infatti, pur modificando in maniera camaleontica l'insieme delle norme sul processo penale, rimane ferma l'esigenza di salvare il Presidente del Consiglio dei ministri. Con questa disciplina transitoria modificata in parte, ma che salva il Presidente del Consiglio - in pratica si dice che il sistema di estinzione si applica ai processi (dunque ove sia stata esercitata l'azione penale) in corso per reati indultabili, per così dire,

del termine di prescrizione qui previsto - due anni - rispetto a quello introdotto a regime - tre anni - è evidentemente un termine *ad personam*.

Fatelo, ma non sfasciate il sistema processuale penale, quello civile e quello contabile.

Signora Presidente, credo che dobbiamo tutti riconoscere, come ha ricordato il relatore, che il Parlamento è in grave ritardo nell'affrontare i problemi sottesi alla Ci sono infatti fattori contingenti, come risulta dalle ultime dichiarazioni del relatore di minoranza, senatore Casson,

che soltanto una corsia privilegiata *contra personam* può garantire la celebrazione dei processi e permettere di arrivare ad una sentenza definitiva per i processi coperti da indulto, che sarebbero raggiunti al 99,9 per cento dalla prescrizione. Ciò, ripeto, se non ci fosse una corsia privilegiata contro una persona, se non ci fosse cioè una scelta predeterminata dell'ufficio giudiziario per arrivare a quel risultato. Allora, se abbiamo tutti consapevolezza di questo dato, possiamo valutare con maggiore calma e tranquillità l'attuazione di un principio costituzionale.

personale; addirittura non si mettono in evidenza - basta leggere i giornali di oggi - gli enormi problemi risolti ieri dal Consiglio dei ministri e le indicazioni forti per un diritto penale più giusto.

Parlo di equilibrio tra le due forti opzioni del nostro ordinamento: la prescrizione del reato e un processo che duri per un tempo ragionevole. Bene, devo riconoscere che dalla sinistra è venuta in questi anni un'attenzione ai problemi posti da questa norma. Io ho difeso personalmente, perché convinto, il progetto Finocchiaro

possono essere rispettati. Luciano Violante nei suoi scritti ha posto varie volte in evidenza come questi tempi sono rispettati in molti uffici giudiziari italiani e in altri no, e tutti siamo consapevoli che la responsabilità affermata dello Stato italiano in relazione alla irragionevole durata dei processi deriva essenzialmente da alcuni uffici giudiziari, e meno da altri. Dobbiamo altrettanto riconoscere che la giurisprudenza della Corte di giustizia europea e quella ormai cristallizzata della Corte suprema di cassazione stabiliscono che la ragionevole durata del processo è di sei anni.

ossia la complessità del processo e la pluralità delle parti processuali. Di ciò siamo tutti consapevoli. La Corte di cassazione continua a condannare lo Stato italiano per la legge Pinto, e la Corte europea esclusivamente perché si superano i sei anni e non vi è complessità del processo o non vi è pluralità delle parti. parti. Non mi si venga allora a dire che non vi è stato uno dibattito parlamentare. Ho molto apprezzato le critiche e gli emendamenti - ne abbiamo parlato in Commissione Colleghi, per cortesia,

differenze rispetto a posizioni soggettive o esclusioni in base ad oggettività del reato.

Qual era il dibattito? Oggi viene previsto dal relatore un tempo di primo grado di tre anni. complessivamente, per i reati meno gravi, un tempo di sei anni e mezzo; ossia non rispetta - vorrei che tutti ne fossimo consapevoli consapevoli - la giurisprudenza che ogni giorno la Corte di cassazione e la Corte europea affermano. Io sono stato, come sapete, sostituto procuratore generale in Cassazione: nei processi, in base alla legge Pinto, sei anni sono troppi, e condanniamo lo Stato italiano. Il relatore ha proposto sei anni e mezzo, e anche su questo trovate da ridire. Nei sei anni e mezzo, scusatemi, ci sono tre anni di primo grado: ma volete tener conto che al primo grado vanno aggiunti i termini delle indagini? Vogliamo tutti dire che se un processo con pena fino a dieci anni non ha raggiunto la sentenza di primo grado dopo tre anni dalla richiesta di rinvio a giudizio, anche conto dei tempi delle indagini preliminari, è destinato a morire per la prescrizione del reato? Ne siamo consapevoli?

che è un termine ampio e che porta complessivamente a sei anni e mezzo il tempo del processo, tradendo la giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte europea. Mi domando per quale motivo

Invece voi sapete che i tempi delle indagini molte volte si allungano a dismisura. L'unico correttivo, grazie al relatore, è quello per il quale, quando sono terminati tutti i termini di proroga delle indagini, si hanno tre mesi di tempo per decidere cosa si intende fare, se rinviare a giudizio o chiedere l'archiviazione. È questa la valenza della norma che viene proposta. quindi legarsi alla norma transitoria per sostenere che vi è un'amnistia strisciante.

cosa è avvenuto dei processi coperti dall'indulto: verificheremo statisticamente quanti sono pervenuti a sentenza definitiva quanti invece sarà dichiarata la prescrizione. Mi domando se la prescrizione del reato sia un principio più forte del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Credo di no. processo. Credo di no. Le proposte di legge formulate nelle passate legislature dall'opposizione non rappresentavano soltanto un'iniziativa dei parlamentari. La scienza giuridica e tutti coloro che si occupavano di esaminare le norme determinate e condizionate dal nuovo articolo 111 della Costituzione si ponevano un problema. Tant'é vero che la commissione ministeriale per la riforma del codice penale, presieduta dall'onorevole Pisapia, e quella per la riforma del codice di procedura penale, presieduta dal professor Riccio (entrambi quindi nominati da Governi dell'opposizione di oggi), entrambe, sia nella riforma del codice penale che in quella del processo penale, all'estinzione dell'azione penale per decorso del tempo.

la regola che ci insegna la Corte costituzionale per cui il principio di obbligatorietà riguarda l'inizio dell'azione penale: anche se i costituzionalisti e gli studiosi di procedura penale tendono a dilatarla, la Corte è rimasta la Corte è rimasta ferma su questi principi. Un minimo di attenzione e di coerenza, allora, dovrebbe portarci oggi ad abbassare il tono del dibattito e dello scontro, che sembra alimentato soltanto dalla preoccupazione di avere forse un'udienza in più in alcuni processi. Badate, a me è dispiaciuto che il Consiglio dei ministri ieri non abbia adottato il decreto-legge; il decreto-legge; io l'avrei proposto. Ne parlavo con alcuni di voi nei corridoi, ed eravamo convinti della necessità di un intervento normativo per garantire parità di trattamento rispetto ai giudici che potranno dare sì la stessa interpretazione ma probabilmente assegnare tempi di riflessione diversi. Eppure si è gridato allo scandalo, come se fosse una norma *ad personam*.

con indipendenza e con coerenza, nel momento in cui ci troviamo ad affrontare la realtà non pensassero all'esistenza di dietrologie o di una volontà di colpire soltanto i processi del Presidente del Consiglio dei ministri. La norma transitoria - dimentichiamo i processi del Presidente del Consiglio dei ministri - è sacrosanta o no? È una norma che avreste approvato nel periodo nel periodo in cui fu presentato il disegno di legge Finocchiaro che prevedeva l'applicazione ai processi in corso? Allora mi domando: vogliamo pensare a realizzare un principio costituzionale o fare una battaglia politica che non ha un risultato concreto dal momento che i tempi di prescrizione del reato sono tali che nessuno potrà toccarli? Vi

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9, 1.35, 1.36 (limitatamente al capoverso 2-*ter*), 1.0.1, 1.0.22 (limitatamente al comma 6), 2.8, 2.11 (limitatamente alle lettere *f)* e 2.200 (limitatamente alla soppressione dell'articolo 4), e 4.200. Esprime parere non ostativo sulle proposte 2.0.4, 2.0.5 e 1.0.21 (testo 2), fermo restando tuttavia che ove uno di tali emendamenti fosse approvato, il parere deve intendersi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sui restanti emendamenti. Esprime infine parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1000/25 e 2.1000/26. Esprime parere non ostativo sulle proposte 1.0.1000/2, 1.0.1000/4, 1.0.1000/5, 1.0.1000/6,

fermo restando tuttavia che ove uno di tali emendamenti fosse approvato, il parere deve intendersi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sui restanti emendamenti. La Commissione osserva infine che le proposte 1.0.1000/15 presentano coperture ultronee. Esprime infine parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

al brutto pasticcio determinatosi in seguito alla insostenibile interpretazione fornita dal Presidente della Commissione giustizia della decisione del Presidente del Senato di rinviare gli emendamenti del relatore in Commissione. Perché insostenibile? È semplice. Perché, ammesso, e naturalmente non concesso, che sia possibile consentire che la maggioranza di una Commissione decida con il voto sulla natura della sede in cui riunirsi per esaminare un affare assegnatole e quindi ammesso, e assolutamente - per quanto ci riguarda - non concesso, che la maggioranza della 2a Commissione permanente potesse decidere con il voto di essere riunita in sede consultiva, risulta dai fatti non dalle mie opinioni che la Commissione giustizia non ha ottemperato neppure agli obblighi derivanti da quella stessa decisione, a mio giudizio - ripeto - illegittima.

Orbene, dov'è, signora Presidente, il parere della Commissione giustizia sull'affare assegnatole, cioè sugli emendamenti del relatore?

deliberante, non era in sede referente, non era in sede redigente e dai fatti risulta che non era in sede consultiva. In quale sede si stava svolgendo allora la riunione della Commissione giustizia che si è tenuta nella giornata di ieri? È chiaro che l'assenza del parere e l'assenza della decisione di mettere in discussione un parere attestano inoppugnabilmente che quella riunione è stata rivolta esclusivamente a vanificare il senso politico e regolamentare della decisione del Presidente del Senato

non passare agli articoli consentirebbe alla maggioranza e al Governo un ripensamento su questa materia. Parliamoci chiaro: tutti sappiamo a cosa serve questo provvedimento i tentativi di nascondere questa verità, che tutti gli italiani normodotati hanno capito, sono patentemente falliti nel corso di queste settimane di discussione.

il Sottosegretario - una legge (nei giorni scorsi si è parlato di decreto) conseguente alla recente sentenza della Corte costituzionale in materia di applicazione dell'articolo 157 del codice di procedura penale. Tra queste tre misure nessuna della quali è da noi condivisa, ma al momento la sostanza non è questa - è certo che l'iniziativa sul cosiddetto processo breve ha sicuri effetti sistemici.

sicuramente gli effetti sistemici del cosiddetto processo breve sono potenzialmente devastanti, mentre non lo sono - se vogliamo dire le cose come stanno - le altre due iniziative di cui si sta discutendo. Decidere ora di non passare agli articoli conseguirebbe quindi due obiettivi: il primo riguarda gli interessi del Paese sul piano politico, poiché si eviterebbe di dare il contributo, forse definitivo, ammesso che già non ci siamo, al processo al processo di sfascio del sistema giustizia del nostro Paese. Il secondo obiettivo è ancora più immediatamente politico perché è in rapporto con le relazioni tra il Popolo della Libertà e il Partito Democratico sul terreno delle riforme costituzionali. Se seguiste la strada degli altri due disegni di legge e non di questo, certamente quel rapporto esile che lega - come dimostrano le due mozioni cosiddette convergenti approvate recentemente dal Senato della Repubblica sul terreno delle riforme costituzionali di iniziativa del PD e del PdL - potrebbe in qualche modo essere ripreso e si potrebbe quindi aprire una prospettiva positiva per il

ieri, il Presidente del Senato ha affermato in quest'Aula di non essere decisamente convinto sull'*iter* che doveva essere seguito in Commissione giustizia dopo il rinvio,

a rinviare nuovamente gli emendamenti del relatore e i subemendamenti in Commissione, perché la Commissione si sarebbe in questo modo sottratta ad un suo obbligo.

garantirà la convocazione della Giunta per il Regolamento per risolvere questo problema. Ma questo problema deve essere risolto prima dei nostri lavori di esame degli emendamenti perché, se poi la Giunta per il Regolamento risolverà il problema dicendo che la Commissione giustizia si è sottratta al suo onere di fase referente, cosa faremo a quel punto? Annulliamo la discussione, rimandiamo gli atti in Commissione giustizia e ricominciamo daccapo? Nel momento in cui viene data la garanzia di investire la Giunta per il Regolamento, ora bisogna farlo e non andando avanti nei lavori! Si risolva questo problema. Se la Commissione giustizia ha operato bene, si vada avanti. Se ha operato male, dovrà dovrà farsi ciò che il Presidente del Senato ha annunciato in Assemblea: non avere nessuna esitazione a rinviare nuovamente gli atti alla Commissione giustizia. Si è detto questo e la tempistica impone di ottenere risposte ora e non domani o la prossima settimana.

ha riferito dell'esistenza di precedenti, in un senso e nell'altro, in ordine all'applicazione dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, chiaramente alludendo a ipotesi nelle quali un provvedimento, rinviato in Commissione ai sensi appunto dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, non era stato sottoposto alla procedura della sede referente, bensì ad altra procedura, dei cui contorni (come spiegato poc'anzi dal senatore Morando) non siamo ancora ben consapevoli. In occasione di questa affermazione del presidente Schifani, ho chiesto quindi agli Uffici di poter disporre di questi precedenti, giacché, dalla ricerca affrettata

stati forniti e mi permetto, quindi, di reiterare questa richiesta, in ragione del fatto che, poiché questo punto dovrà andare all'esame della Giunta del Regolamento, sarebbe bene avere una compiuta casistica delle diverse prassi adottate dal Senato, se di diverse prassi possiamo parlare.

Stiamo esaminando in Aula un testo totalmente diverso da quello che la Commissione per circa un mese ha studiato, istruito ed approfondito con audizioni, con una valutazione in ordine all'impatto

il relatore e la maggioranza in via prudenziale a far approvare un emendamento con una clausola - chiamiamola in questo modo - di salvaguardia finanziaria ai sensi dell'articolo 81, ancorché debole dal nostro punto di vista. a confrontarci con un provvedimento che cambia sostanzialmente una serie di regole, che introduce peraltro nuovi istituti con riferimento al giudizio contabile, che cambia il livello di applicazione e di impatto della normativa rispetto ai giudizi in corso.

un forte impatto non solo sull'intero sistema giudiziario e sull'ordinamento processuale, ma anche sui giudizi davanti alla Corte dei conti, sui giudizi amministrativi e su quelli civili. Tutto questo ovviamente determina una serie di conseguenze che non siamo nelle condizioni di poter Ripeterò fino alla noia - sarò stancante, signora Presidente, ma mi permetto di ricordarlo - che, quando quest'Aula ha stralciato alcune norme del pacchetto sicurezza e ha prodotto un esame parlamentare di un complesso di norme scollegato dal decreto-legge e nell'ambito di un disegno di legge ordinario riguardante un complesso di norme a cui pure l'opposizione ha concorso (mi riferisco ad esempio alle norme antimafia e così via), in quella circostanza fu inserita una serie di disposizioni eterogenee che non avevano né una loro coerenza intima intima né una loro connessione funzionale rispetto all'originario complesso di norme proposte dalla maggioranza. Rispetto a questo il Capo dello Stato è stato costretto ad intervenire con una lettera indirizzata al Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio, al Ministro dell'interno

all'ultimo minuto con un provvedimento totalmente diverso, nuovo, rispetto al quale non siamo neanche nelle condizioni di proporre alcuna forma di modifica. Il fatto ancor più grave che determina una forzatura ed una innovazione inaccettabile sul piano del procedimento legislativo è che tutto il

solo ed esclusivamente al maxiemendamento presentato dal relatore. Quindi, in realtà, ci troviamo di fronte a un triplice problema ed il primo è quello dell'esame ed approvazione di un provvedimento in Commissione diverso da quello che voteremo in Aula. Inoltre, rispetto alle materie che sono oggetto di confronto parlamentare, poiché è chiaro che ci concentreremo solo ed esclusivamente sull'attività relativa agli emendamenti e ai subemendamenti che sono stati presentati, anche l'attività legislativa sarà circoscritta e la materia su cui ci ci concentreremo sarà quella dettata dal maxiemendamento del relatore. Credo che tutto questo non ci metta nelle condizioni di fare una valutazione serena e obiettiva del provvedimento in esame. Per queste ragioni, riteniamo sia opportuno non passare all'esame degli articoli e riprendere un ragionamento sulla ragionevole durata del processo che riteniamo sia utile al Paese, ma la ragionevole durata del processo è una cosa diversa da ciò che stiamo facendo in

di aver fornito al senatore Legnini i documenti ed i precedenti. Nel caso di specie, la Commissione ha deciso con un voto come procedere. Ricordo altresì che ieri il presidente Schifani ha affermato di riservarsi di investire la Giunta per il Regolamento per riesaminare a fondo la questione. La Presidenza non può che confermare questa decisione.

abbiamo assistito ad una relazione imbarazzata, cui è seguita una replica ancora più imbarazzata, e ad un intervento giuridicamente incomprensibile fatto dal sottosegretario Caliendo. Ci si dice: dimentichiamo il fatto contingente, ossia la necessità di dover approvare questo disegno

ragioniamo sulla bontà di questo provvedimento a prescindere dal fatto che c'è un motivo contingente che lo impone.

un'opzione paragonabile ad un decreto con cui si decide che una FIAT 500 possa partecipare ad un gran premio per il campionato mondiale delle altre

afflitto da patologie e da tempi sicuramente notevoli lo facciamo diventare veloce,

si conclude entro il termine previsto muore. Questa non è una norma che accelera i processi! È una norma che ne decreta la morte, processi per reati puniti fino a dieci anni meno un giorno, cioè reati gravi. Migliaia di delinquenti verranno graziati da una norma che avrà un effetto permanente. Con l'indulto, che era stabilito nella misura sino a tre anni della pena, sono usciti dal carcere 27.000-28.000 condannati, con questa norma reati puniti con pene sino a dieci anni meno un giorno vedranno la morte e migliaia

verranno rimessi in libertà, se in carcere, o verranno di fatto amnistiati. Questa non è un'amnistia per reati fino a quattro anni, come nella storia è sempre accaduto, ma per reati sino a dieci anni. Ciò non era mai accaduto nel nostro Paese: si introduce un'amnistia permanente per reati sino a dieci anni: una cosa del genere non era mai accaduta ed è contraria a qualsiasi

E voi dite che questa è una legge fatta nell'interesse degli italiani?

deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari, quindi il termine previsto dall'articolo 407 Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi precedenti; allora i tre anni iniziano a decorrere dai due anni e tre mesi, termine delle indagini preliminari: tre mesi aggiunti.

rispettare. Vogliamo lavorare per migliorare il sistema giustizia; ecco perché il nostro emendamento

che alla prima udienza bisogna risolvere tutti i problemi che riguardano le questioni preliminari e fissare il programma del processo vincolante per le parti, cioè le udienze Questo è quello che proponiamo: si deve intervenire sul processo, ma obbligando le parti della prima udienza tutto il programma del processo con la calendarizzazione delle testimonianze e delle altre prove da assumere, con date

che mi pare più agevole, più semplice da intraprendere e quindi più utile alla collettività. È prevista l'introduzione della domanda anche direttamente da parte dall'interessato. Si stabilisce una fase che si potrebbe definire sostanzialmente "cartolare" in forza della quale l'interessato può avanzare la domanda alla competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, vale a dire la corte d'appello del distretto vicino a quello in cui si celebrò il processo nel cui ambito è stata lamentata la violazione che poi dà luogo alla richiesta di indennizzo. La domanda, una volta presentata alla corte d'appello, viene poi delegata ad un consigliere. Non è più la corte nella sua interezza, e dunque con la complessità oggettiva che la collegialità comporta, a giudicare di un fatto che ha

Quindi, sarà il consigliere delegato ad occuparsene, a valutare entro un tempo assolutamente ragionevole se sussistano

la ragione per la quale viene accolta o meno la domanda del ricorrente. Avverso questa pronunzia,

collegialmente costituitasi. Quindi, nell'ambito della corte d'appello si esaurirebbe la fase di merito della richiesta la fase di merito della richiesta avanzata per violazione della legge Pinto e tutto ciò renderebbe molto più semplice l'*iter*, tenuto conto che la prima la prima richiesta non avrebbe neanche necessità del conforto particolare di un'assistenza professionale. L'assistenza professionale è obbligatoria soltanto nel momento in cui si dà luogo all'impugnazione. Le violazioni di legge naturalmente sarebbero censurate nella sede di legittimità, nel rispetto rigoroso dell'articolo 111 della Costituzione. A me è parso che questa formula sia più agevole e più semplice; una formula che interviene in maniera più opportuna sulle esigenze della collettività: il cittadino si rivolge direttamente al suo giudice per ottenere giustizia. Ritengo che non vi è ragione di censurare, com'è stato fatto,

di rivolgere un invito al relatore e al rappresentante del Governo. Per un provvedimento così importante, per il quale, peraltro, come abbiamo ampiamente dibattuto ieri e oggi, non c'è stata da parte della Commissione di merito una valutazione su parti

richiamo ad una norma regolamentare che, ripeto, preclude la possibilità di esprimere un parere sintetico in blocco su tutti gli emendamenti. Il ministro, senatore Calderoli, a suo tempo, su questa materia ci intrattenne in più occasioni, se non ricordo male.

ai sensi dell'articolo 148 del codice di procedura penale. Devo prendere atto che il Governo ha presentato un decreto-legge per la razionalizzazione del processo in cui recepisce le nostre proposte.

Signora Presidente, come spesso accade trattando di questioni di vitale importanza, non c'è tempo; i tempi sono contingentati, abbiamo pochi minuti. Dovremmo dire tanto, ma io scelgo di fare un intervento che spero possa essere puntuale, e spero soprattutto che qualcuno dei colleghi della maggioranza, violando l'ordine di chiudere l'audio, ascolti quello che sto per dire. Questa è una legge dannosa per il Paese. È una legge che contiene menzogne dall'inizio alla fine. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di correggerla, offrendo un sincero apporto, presentando emendamenti che non sono di tipo ostruzionistico, ma sono ragionevoli, anzi sarebbero indispensabili per dare dignità di legge a questo atto che voi state per imporre.

In questo parere è scritto chiaramente quanto segue: «si invita a valutare l'impatto che la rigidità dei termini di durata può determinare sull'ordinamento e a considerare (...) l'introduzione di alcune clausole di flessibilità». Vuol dire che questo disegno di legge così com'è non va. Inoltre: «si segnala l'opportunità di valutare, in ragione dell'entità dei processi interessati, la praticabilità della corsia preferenziale per i processi nei quali sia stata presentata istanza di accelerazione dopo il trasferimento dell'azione in sede civile». Vuol dire che ci sarà un ingolfamento, cioè un effetto diametralmente opposto a quello che la legge dichiara di volere perseguire. Terza osservazione: «si richiama (...) l'opportunità di integrare il provvedimento con misure volte ad accelerare lo svolgimento dei processi, individuando interventi specifici e immediati che assicurino una riduzione» effettiva dei tempi del processo. Questo documento importantissimo, che la Commissione giustizia ha totalmente ignorato, afferma che il parere favorevole è sostanzialmente subordinato all'accoglimento di tutti gli emendamenti e lo ribadisce in termini chiari in finale

dirette a renderlo più celere, e la garanzia di durata certa». Voi avete sostenuto, attraverso l'intervento sia del senatore Valentino, sia del rappresentante del Governo, che questa è una legge positiva. Avete una forza e un'impudenza che veramente meraviglia l'uomo comune. Sostenete falsità assumendo di volere soddisfare esigenze del Paese e varate una legge che produrrà soltanto danni. Avviandomi alla conclusione, voglio proporvi una semplice addizione, un'operazione aritmetica. Abbiamo proposto il sistema informatizzato; è un sistema che abbiamo studiato e prodotto nella scorsa legislatura e che vi abbiamo offerto lealmente per la sua attuazione. Vi ostinate a svicolare e non lo volete attuare perché sarebbe uno strumento importantissimo per rendere effettivamente più brevi i processi. Questo è il primo addendo. Il secondo riguarda 2.800 cancellieri da assumere, perché le cancellerie sono paralizzate. È questa una delle ragioni per cui i processi sono lunghi. Perché

2.800 cancellieri? Le cancellerie sono paralizzate e voi stabilite per legge ciò che non può essere fatto in pratica. Il terzo concerne l'ufficio per il processo. È detto con chiarezza nel nostro disegno di legge e nel relativo emendamento cos'è l'ufficio per il processo: uno strumento per non dare alibi neppure a quei magistrati (una minima percentuale) che non intendono lavorare o che non riescono a lavorare. Ancora: nuova organizzazione delle cancellerie e ripresa della riforma del processo penale, o del penale, che è già in atto in atto presso la nostra Commissione e che avete bloccato. In fondo a questa addizione c'è un segnetto che dice uguale: uguale processo breve. Due domande, allora, e chiudo. perché non avete accettato gli emendamenti che vi abbiamo proposto, che avrebbero dato dignità ed efficacia a questa legge, e sostenete ancora oggi, con un'impudenza veramente eccezionale, che questa è una legge positiva che va applicata? varerete voi, assumendovi questa responsabilità storica. Seconda e ultima domanda: se veramente non è una legge censurabilissima, anche dal punto di vista della sua natura di legge *ad personam*, perché non abolite seduta stante - relatore, proponga di revocarla! - la norma transitoria? A quel punto noi saremmo molto ma molto più comprensivi e il Paese capirebbe che finalmente non mentite ma volete fare qualcosa di utile.

in relazione a richiami a disegni di legge del centrosinistra di precedenti legislature, in particolare a quelli del senatore Fassone e del senatore Brutti. Ora, quei disegni di legge in materia di prescrizione, e soprattutto il disegno di legge presentato in questa legislatura dal Partito Democratico, sono alcune proposte che vengono inserite all'interno di un pacchetto di modifiche

danno perfettamente contezza del fatto che il Partito Democratico ritiene indispensabile intervenire con un insieme di misure sulla macchina della giustizia.

un sistema sinergico di prescrizione sostanziale e processuale del reato: il tempo trascorso dal momento di commissione del reato rileva anche in funzione degli atti processuali realizzati e dunque delle modalità di esercizio dell'azione penale. La disciplina della prescrizione proposta dal Partito Democratico si orienta su alcune direttive principali. Innanzi tutto,

si sia manifestato tramite l'esercizio dell'azione penale. In secondo luogo, i termini del primo tipo di meccanismo prescrizionale devono essere parametrati in funzione della gravità del reato, valutato sulla base della pena edittale, tenendo conto delle eterogenee comminatorie edittali presenti nel nostro ordinamento. Inoltre, vengono previste cause di sospensione della prescrizione cosiddetta processuale,

o l'espletamento di rogatorie internazionali che, come noto, riguardano spesso anche l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri. All'esito di queste considerazioni, il disegno di legge del Partito Democratico, quanto

Per quanto concerne la decorrenza dei termini di prescrizione, la proposta del Partito Democratico prevede che, ove sia stata esercitata l'azione penale entro i termini indicati dal codice di rito processuale

bisogna prenderne atto e onestà intellettuale vorrebbe che questa speciosa e strumentale polemica, sollevata anche stamani, finisse. Invito, dunque, la maggioranza ed il Governo a non coprire le loro magagne e i loro favori a ben determinate persone

provvedimento che regola la procedura della cosiddetta legge Pinto in maniera differente e pone presupposti di fondo perché i provvedimenti giudiziari vengano considerati ed emessi in tempi ragionevoli.

incrementare significativamente le richieste di equa riparazione rispetto alla situazione attuale. Tutto questo si riflette sulla giustizia civile, che viene ad essere così indebolita, mentre essa è un presupposto essenziale per la nostra democrazia e per l'economia del Paese. Mi riporto per questo alla questione sospensiva da me presentata,

come messo in luce da recenti studi economici - finisce con l'avere un effetto negativo sul mercato del credito, sullo sviluppo finanziario, sul credito commerciale, sulla natalità e sulla dimensione delle imprese

Questa è la ragione per la quale proponiamo mezzi di velocizzazione del processo e, tra questi, innanzitutto, quello che prevede la non offensività del fatto e quindi una pronunzia di non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato, non integra più una fattispecie penale, laddove si tratti di offese che non abbiano il carattere di rilevanza. Si tratta di salvaguardare in questo modo l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale che è ragione di garanzia ed eguaglianza, trovando però rimedi che possano essere attuati subito.

gli avvocati penalisti, che hanno richiamato l'attenzione del Governo e della maggioranza sul punto che non si può procedere ad una riforma del processo penale e del processo civile - che si realizza attraverso la rielaborazione della legge Pinto - se non si tiene conto che nel nostro ordinamento non possono essere inseriti reati che non hanno rilevanza penale, come invece è accaduto, e che spostano l'offensività del fatto sulla qualità dell'autore del reato: mi riferisco al reato di immigrazione clandestina. Se così è, potremmo subito concordare una misura, che mi pareva che il relatore Valentino avesse accolto anche positivamente durante il nostro dibattito in Commissione; non comprendo perché questa misura che, oltretutto, è

creando così una deflazione del processo penale, in maniera tale da dare più spazio alla possibilità per i cittadini di ottenere giustizia.

la lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 2 della legge Pinto e, quindi, di escludere la possibilità

da un processo lungo, più che quello patrimoniale, sia proprio il danno di immagine. Non capisco la ragione per la quale si debba sopprimere la disposizione che tutela e garantisce la risarcibilità del danno di immagine derivante dall'irragionevole durata del processo. Questa mi sembra una contraddizione perché, comunque, il ristoro economico, per quanto possa essere consistente, non sarà mai equivalente, come è noto,

Se vi vuole realmente mettere mano con serietà alla legge Pinto, io non comprendo la ragione per la quale si vuole sopprimere la disposizione che consente la risarcibilità del danno non patrimoniale.

Poretti. L'individuazione dell'assunzione della qualità di imputato come inizio di decorrenza del termine previsto per la ragionevole durata del processo penale, secondo questo emendamento e secondo noi, è in contrasto con l'articolo 111 della Costituzione, il quale ricomprende nel concetto di processo anche la fase delle indagini, almeno nel momento in cui l'interessato abbia avuto la percezione della loro esistenza.

per tutta la durata del processo - così come ha detto sempre la Corte di giustizia europea e senza tenere conto, tra l'altro, degli degli elementi che possono giustificare la lunghezza del processo - addirittura in due anni per il primo grado che - badate bene - non vanno contati dal momento della citazione o dall'inizio del giudizio di primo grado,

che dà luogo al risarcimento dei danni a norma della legge Pinto, complessivamente

processi puniti con pena massima inferiore a dieci anni. Poi, però, arriviamo a tempi abbastanza lunghi quando la pena massima supera i dieci anni, in quanto si stabilisce

se il diritto al risarcimento dei danni rimane quello stabilito nell'articolo 1, possiamo mantenere veramente in piedi il capoverso e dare la possibilità a tutti gli imputati di reati più gravi, per i quali è stabilito un termine più lungo, che quindi

quanti saranno i risarcimenti dei danni da pagare. Ci vorrà molto perché la criminalità organizzata si accorga di questa incongruenza e chieda sistematicamente l'accelerazione dei processi e, quindi,

stata formulata, soprattutto in relazione al fatto che si approverà quasi certamente il maxiemendamento presentato dal relatore?

è stato capofila di un progetto europeo sulla ragionevole durata del processo appreso che i tempi medi e i tempi che segnano, per un processo civile, la ragionevole durata del giudizio di primo grado prevedono tre anni. anni. Credo che, se vogliamo fare realmente un lavoro utile a stimolare la magistratura a lavorare in termini di maggiore efficienza, senza per questo determinare una tagliola automatica che precostituisce il diritto all'equo indennizzo per centinaia di migliaia di giudizi, con una sovraesposizione finanziaria del bilancio del Ministero della giustizia che nessuno è nelle condizioni di poter quantificare, dovremmo in qualche modo cercare di cambiare questo meccanismo. La proposta contenuta nell'emendamento 1.24 è stata quella di definire in tre anni la ragionevole durata del giudizio di primo grado, in due anni quello d'appello ed in un anno quello di cassazione, fermo restando che, anche ai fini della ragionevole durata del giudizio di rinvio a seguito di decisione della Suprema corte, non si può predeterminare un tempo rigido, il tempo della ragionevole durata del giudizio di rinvio è determinato dalla natura del giudizio a cui si rinvia, se di primo grado o se d'appello e così via. Allora, se così è, ritengo che buon senso vorrebbe

Questo anche per un'altra ragione, che non è solo quella di salvaguardare l'erario da una sovraesposizione finanziaria dovuta alla circostanza che il diritto all'equo indennizzo scatta automaticamente in virtù del decorso del tempo, senza verificare la complessità o meno del giudizio, ma in del fatto che voi state introducendo una norma che, ad esempio, differenzia per il giudizio contabile la ragionevole durata in ragione dell'importo presunto del danno che si contesta al convenuto: presuntivamente un danno erariale di 200.000 o 300.000 euro - ora non ricordo - dura due anni, se è superiore a 300.000 euro dura tre anni. Non credo che un giudizio

è complesso in ragione delle parti convenute, della questione giuridica che si tratta, delle amministrazioni che sono coinvolte, del tipo di legislazione finanziaria e contabile che è presa in considerazione, della natura dei provvedimenti che vengono adottati e così via. Allora è evidente che fissare una soglia temporale in maniera così acritica e rigida, come voi state facendo, serve solo a scalzare i giudizi senza che a questo corrisponda alcun tipo di effettivo ristoro per il cittadino che si trova ingiustamente danneggiato dall'assenza di giustizia. Queste sono le ragioni per le quali riteniamo che una proposta di questo tipo possa essere di buon senso, senso, in linea con le esigenze di fare la ragionevole durata del processo, se volete fare la ragionevole durata del processo; se volete fare un'altra cosa, è evidente che il mio emendamento è poco attuale. Chiediamo la votazione

Presidente, stamane, prima con un intervento del senatore Morando e del senatore Li Gotti e poi con un intervento mio, avevamo sottolineato che che l'esame da parte della Commissione giustizia del testo del relatore che era stato inviato era stato non coerente rispetto al nostro Regolamento e, più complessivamente, rispetto ai principi che devono reggere il funzionamento del Senato, a cominciare da quello che riguarda il diritto delle opposizioni di vedere discussi i testi. Ho ricordato nel mio intervento come lei ieri avesse sottolineato che la prassi

disposizione della Commissione giustizia a decidere di seguire uno dei filoni interpretativi e cioè quello che riguardava il fatto che nella Commissione non si dovesse procedere secondo le regole che governano il procedimento in sede referente. Stamattina il senatore Morando ha evidenziato come la Commissione non avesse agito neanche nell'altro possibile modo, cioè quello regolato dalle disposizioni in materia delle competenze della Commissione in sede consultiva, ed io mi sono permessa di reiterare una richiesta che avevo già avanzato nella giornata di ieri agli Uffici perché potessi valutare non soltanto i precedenti favorevoli alla nostra tesi, e di cui ieri avevo dato ragione in questa Aula, ma anche gli altri a cui lei aveva fatto riferimento per dare atto di una controversa prassi. Nel pomeriggio di ieri - l'ho appreso solo successivamente al mio intervento - al senatore Legnini era stato fornito dagli Uffici della Presidenza un precedente che, secondo la prospettazione che ne veniva data, appunto, dagli Uffici della Presidenza, militava a favore della scelta operata ieri dalla Commissione giustizia. Abbiamo valutato questo precedente, Presidente, e questo caso mai conferma, piuttosto che smentire, le nostre posizioni. Si tratta di una vicenda che risale al giugno 2000, presidenza Mancino, e che intervenne nel corso della discussione di un provvedimento in materia di fecondazione assistita, se non ricordo male. In tale contesto, poiché un emendamento presentato, a parere della Presidenza, poteva avere un'incidenza devastante sul testo del provvedimento e comunque al fine di valutare quali potessero essere sul rimanente testo ancora da esaminare le conseguenze dell'approvazione di quel famoso emendamento, con un mandato preciso con un mandato preciso che faceva riferimento alle prerogative in materia di procedimento in sede consultiva, il provvedimento veniva rimesso dal Presidente del Senato alla Commissione.

direzione delle obiezioni che abbiamo più volte formulato e sulle quali mi permetto di insistere. questo precedente che le è stato trasmesso si espone a varie interpretazioni, e le potrei dire che comunque la Commissione ha concluso i propri lavori senza votare gli emendamenti.

Presidente, credo che, anche a proposito dell'articolo 1, si debba evidenziare un aspetto di grande importanza che è stato trascurato e forse ignorato fino a questo momento. Infatti, l'approvazione del disegno di legge

particolare, un articolo 3-*ter* che sancisce una presunzione *iuris tantum* di non irragionevole durata dei procedimenti giurisdizionali dinanzi a qualsiasi giudice, sia ordinario che speciale. (si parla di corsia preferenziale) in sostanza determinerà un incremento rilevante dell'attività del giudice civile, che è chiamato a determinare il danno e a risarcire delle spese delle spese un numero crescente, indefinito e indefinibile, di parti offese. Questo sistema non potrà che incidere sulle casse dello Stato. L'articolo 2 del disegno di legge, nell'introdurre nel nuovo codice di rito penale una peculiare ipotesi di improcedibilità causa sopravvenuta, prevede conseguentemente... Signor Presidente, il Governo e il relatore sono disinteressati, come sempre. *(PD)*. ...una disciplina speciale per il trasferimento in sede civile dell'azione giù intentata. Insomma, si interrompono i processi penali e si aumenta a dismisura il numero dei processi civili senza - lo evidenzio

Il potente di turno si fa "cucire" la legge che gli serve! Ora siamo arrivati al condono per il danno erariale

di sei dipendenti dell'ufficio stampa, impiegati, a partire dal 2006, con lo stipendio che negli enti pubblici a norma di legge è riservato ai dirigenti e senza averne i requisiti, a cominciare dalla laurea. Questa è una norma fatta

credo che anche questo articolo ci renda impopolari nella maniera più assoluta. In sostanza, si vuole sottrarre il potere politico anche al controllo di tipo contabile.

può essere presentata dall'interessato l'istanza di fissazione dell'udienza, cioè non è vero che vi può essere una durata illimitata nei processi contabili.

un'istanza che obbliga a fissare la discussione del processo contabile entro 90 giorni. Non solo, ma che l'udienza sia fissata e tenuta effettivamente entro i 90 giorni è lasciato proprio alla responsabilità del presidente. Ebbene, se così

è chiaro che il *dominus* della durata del giudizio di conto è il pubblico ministero presso la Corte dei conti, il quale quantificherà il danno nella contestazione dell'addebito che fa al convenuto. Se contesta un danno erariale - poco importa poi quale sarà la condanna finale che è al di sotto dei 300.000 euro, il giudizio durerà due anni; se è al di sopra di questo importo, il giudizio durerà tre anni. È evidente che questa è una castroneria. È evidente che porta all'effetto opposto,

sbagliata. Come è altresì sbagliata l'idea di non consentire non al pubblico ministero presso la Corte dei conti, ma al collegio chiamato a giudicare sulla responsabilità erariale, di disporre l'unico mezzo di prova che ha nel giudizio contabile per accertare la veridicità dei fatti e quindi controbilanciare, contraddire le contestazioni del pubblico ministero, ossia le ordinanze istruttorie. poiché per fare un'ordinanza istruttoria occorrono sei mesi di esecuzione, è chiaro che, a fronte di un giudizio che dura - altrimenti si estingue - due o tre anni, nessuno disporrà questo mezzo istruttorio. E poiché l'ordinanza istruttoria è uno strumento

Lega. Non venite poi a dire che paga Pantalone. Non venite più a romperci le scatole - mi scusi il termine, Presidente - con tutte le chiacchiere su chi paga, sulla trasparenza, sui cittadini, sul federalismo fiscale. Questa, infatti, è l'ultima pietra miliare nella demolizione della tutela dei cittadini nei confronti di quegli amministratori che sperperano il danaro pubblico. L'unico soggetto che può giudicare del danno erariale è la Corte dei conti, la quale con detta norma, oltre a quelle che avete già approvato, va in vacanza. Faremo una bella campagna elettorale su questo punto, ma almeno tacete e non dite più che è necessaria la trasparenza, perché Pantalone se ne è andato in vacanza.

È altamente probabile che si verifichi la prima ipotesi, altrimenti non ci sarebbe ragione per introdurre una norma di questo tipo, tanto più all'esito della riflessione che ha portato alla presentazione degli emendamenti da parte del relatore. questa mattina avevo contestato la decisione del relatore e del rappresentante del Governo di esprimere pareri in forma sintetica, nel senso che - come abbiamo ascoltato

della effettiva portata di questa norma, sia *de futuro* sia sui processi in corso, non abbiamo potuto discutere in alcuna sede: non abbiamo potuto discutere nella Commissione di merito, a causa della nota decisione di non esaminare e votare gli emendamenti del relatore in quella sede; non se ne può discutere in Aula, perché non abbiamo ascoltato neanche mezza parola dal relatore e dal Governo su una delle norme più impattanti sulla responsabilità degli amministratori pubblici, dei soggetti investiti di funzione pubblica, e anche sulle casse dello Stato. Infatti, si potrebbe si potrebbe verificare (anzi, si verificherà certamente) che l'estinzione di centinaia di migliaia o di decine di migliaia di processi pendenti davanti alla Corte dei conti determinerà

per rispetto della nostra funzione. Cosa state votando? Cosa andrete a votare? Chi sarà il beneficiario di questa norma? Qual è il rapporto, signor Presidente, tra l'emendamento 1.0.1002 e la disciplina transitoria che

si applicano anche ai giudizi in corso, purché siano trascorsi cinque anni dall'avvio dell'azione risarcitoria

fino a mercoledì prossimo? Almeno discutiamo di questa materia delicatissima, che coinvolge molti interessi.

a votare. Almeno dateci il tempo di valutarlo anche in rapporto all'emendamento che reca le disposizioni transitorie a cui mi riferivo in È una questione molto delicata e molto importante, signor Presidente. La prego di vagliare la richiesta nel modo che l'importanza del tema merita. Presidente, avevo chiesto di parlare esclusivamente perché all'inizio dell'intervento il senatore Legnini aveva prospettato l'ipotesi che l'articolo 1-*quater*

Certo, è un'altra disciplina. Questa disciplina non si applica ai processi in corso. È l'altra normativa.

di tutti i processi, di tutti i procedimenti, ogni qual volta sussista la pretesa punitiva o risarcitoria dello Stato si è ipotizzata una sanzione di natura processuale, nel caso tale richiesta non fosse formulata entro termini coerenti con i principi costituzionali. Naturalmente, le norme che contengono sanzioni processuali non valgono per i giudizi civili e amministrativi dove l'eventuale sanzione è soltanto la possibilità di indennizzo prevista dalla legge Pinto. Non si coglie un'alterazione del sistema, ma anzi una coerenza con l'impianto che si intende stabilire con la nuova norma. Naturalmente,

Presidente, è contrario all'accantonamento perché sia per i processi penali, come per questo processo contabile, le norme che vengono introdotte rappresentano un modello organizzativo a cui i capi degli uffici si devono attenere nell'organizzazione. I tempi previsti sono già lunghi e mi pare possano essere rispettati;

il termine, la «tagliola», è di cinque anni dal deposito dell'atto di citazione presso la segreteria della sezione giurisdizionale, ma noi sappiamo bene - e credo che lo sappiamo tutti che i giudizi contabili di responsabilità in primo grado durano mediamente tre anni. Questa, quindi, è una norma che può servire in qualche modo a un effetto deflattivo del carico di lavoro presso le sezioni giurisdizionali di primo grado con riferimento a quei processi che, rispetto alla media, hanno una durata eccessivamente superiore. mi si passi l'espressione (non vorrei essere frainteso politicamente): «che c'azzecca» l'applicazione indiscriminata di questa disciplina ai processi in corso in fase di appello, indipendentemente dalla durata degli stessi? Signor Presidente, l'intervento del Governo del Governo richiede una puntualizzazione, in quanto ha detto cosa non rispondente a realtà. I casi disciplinati sono di tre tipi, fra cui il procedimento per il quale è stata depositata la richiesta di citazione che non si è concluso nei cinque anni, quindi pendente. Si tratta dell'ultimo inciso della norma transitoria,

le nuove norme si applicano «nella» fase di appello. Non c'è scritto che si applicano «alla» fase di appello, ossia che riguardano i procedimenti di appello, ma che si applicano «nella» fase di appello agli altri casi, ossia qualora un procedimento di primo grado si sia concluso in due anni ed un giorno.

non «alla» fase di appello. Quindi, «nella» fase di appello si deve valutare la durata del tempo della fase di primo grado, qualora il giudizio si sia concluso.

È solo questo: la fase transitoria è soltanto per i cinque anni; ora, se volete continuare a fare questioni, si tratta di stabilire che nella fase di appello non ha più senso mantenere un termine diverso, perché se c'è il primo grado ora, quando si arriva nella fase di appello sarà di due anni, proprio per quel motivo organizzatorio.

«Negli altri casi si applicano alla fase d'appello».

abbiamo accertato che c'è la norma che si applica ai giudizi contabili in corso e che certamente queste norme sull'estinzione si applicano ai giudizi d'appello, però su questo né il relatore né il Governo ci hanno dato una risposta; abbiamo accertato che esse si applicano ai giudizi di primo grado se hanno una durata superiore ai cinque anni dal deposito della citazione in giudizio presso la segreteria della sezione giurisdizionale. Manca anche la terza ipotesi, che pongo, sperando di ricevere almeno su questo una risposta: cosa succede per tutti quei procedimenti iniziati con le contestazioni del pubblico ministero presso la Corte dei conti, quando questi non abbia ancora provveduto al deposito della citazione

accontentarsi della precisazione in termini di interpretazione in forza della quale riguarda solo il grado di appello, è un problema suo; per quanto ci riguarda, le questioni che abbiamo sollevato restano tutte là.

al fine di riproporre tali modifiche in un nuovo emendamento, che tengano conto del dibattito, nei limiti della compatibilità e dell'ammissibilità delle obiezioni con il contesto normativo.

dinanzi ad una ipotesi di delega al Governo perché vari il sistema integrato giudiziario informatizzato, laddove poi non si bada alla mancanza gravissima di copertura per tutto ciò che accadrà a seguito dell'approvazione di questo disegno di legge. Il Presidente della 5a Commissione farebbe bene a spiegarmi come è possibile che sia sfuggita la mancanza di copertura, e quindi la violazione dell'articolo 81 della Costituzione, dinanzi ad un disegno di legge che prevede automaticamente il riversarsi di un numero indefinito ed indefinibile di cause civili, che automaticamente porteranno alla condanna dello Stato perché per legge è stato violato

ad accorciare i tempi del processo. Perché la maggioranza si ostina a dire di no anche ad emendamenti del genere, che indubbiamente darebbero la possibilità di ridurre un tantino i tempi del processo? Perché si continua a dire di O non vi state rendendo conto della gravità di ciò che sta accadendo in quest'Aula oppure non riesco a comprendere le ragioni per cui interventi correttivi agevolatori

di delega al Governo finalizzata a trovare la possibilità di attuare in tempi brevi un sistema integrato giudiziario informatizzato che è stato da noi studiato e predisposto nella scorsa legislatura e che voi ancora non attuate perché non avete veramente in nessuna considerazione gli interessi reali

i quali normalmente lavorano dalle ore 8 alle ore 14, ovvero quando di solito lavorano anche tutti quelli cui deve essere portata la notificazione.

idea è che la prima notificazione all'imputato venga fatta a mani proprie e non per finzioni.

perché non c'è certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo che si

fare in modo che vi sia assoluta certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'esistenza del processo a suo carico, con la notificazione a mani proprie. È una questione importantissima, e mi dispiace che si sorvoli in questo modo.

un'altra delle ragioni per cui veniamo condannati (perché è una finzione di conoscenza quella del decreto di irreperibilità che viene completamente eliminato e sostituito da questa sospensione del processo quando l'imputato non è più reperibile), ma acceleriamo anche notevolmente i tempi dei processi. Infatti, quando notifichiamo a mani proprie diciamo all'imputato: «Guarda che hai un difensore d'ufficio, che è questa persona, con questo indirizzo, questa *e-mail* e questo numero di telefono; le successive notifiche saranno fatte presso questo difensore o presso il difensore di fiducia che hai nominato». Si determina in tal modo un'accelerazione dei tempi e un'assoluta esclusione di qualsiasi nullità della notifica che è senza paragoni.

dell'Assemblea su quanto sia importante modificare il sistema delle notificazioni, tant'è vero che anche voi nel disegno di legge n. 1440 avete stabilito una delega al Governo in materia:

Qui non si spende una lira per fare questa modifica al codice: al contrario, si fanno risparmiare allo Stato italiano milioni e milioni di euro per condanne a risarcimento danni che subisce in continuazione dalla Corte europea, o comunque per l'applicazione della legge Pinto. Se vogliamo discutere seriamente del processo breve e se vogliamo veramente

poco considerevole di soldi: basta guardare le somme pagate negli ultimi anni dallo Stato a titolo di risarcimento per la legge Pinto e le domande di risarcimento danni che sono state avanzate.

maggioranza non c'è nessuna volontà di ridurre radicalmente i tempi dei processi e di far risparmiare allo Stato italiano le somme ingenti che paga per il risarcimento dei danni.